La ragione eevidente: attendere l’arrivo dei colleghi della maggioranza. Questa continua tentazione di adattare le regole alle esigenze della maggioranza – ieri ne abbiamo avuto un’ulteriore dimostrazione – e assolutamente inaccettabile. Ho inteso sottolinearlo, perche´ non possiamo tollerare la continua violazione delle regole che sovrintendono ai lavori del Senato.

parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 4.

Abbiamo giaosservato come nella formulazione della norma ci sia una sorta di ideologia presidenzialista, per cui nell’elenco degli organi il rettore viene prima del senato accademico. A rigor di logica dovrebbe venire prima il senato accademico e poi il rettore. In questo elenco, in una forma incrociata, esistono due presidenzialismi: il rettore e il direttore generale.

di una filosofia aziendalistica a danno dell’autonomia della comunita scientifica.

altresı dire che l’Italia dei Valori ritiene il provvedimento un inutile braccio di ferro che il Governo sta imponendo al Parlamento e al Paese, pur non rappresentando la maggioranza degli italiani. Un vero eproprio atto di forza che il centrodestra, incurante del clima di particolare tensione che inquina la riforma, causato anche dall’arroganza del ministro Gelmini e della sua coalizione, che non hanno inteso ascoltare ne´ gli studenti, ne´ i ricercatori, ne´ i precari, che vengono sacrificati da una legge sbagliata. Massacrare la ricerca e l’universitapubblica e fuori da ogni logica e va contro l’interesse del Paese. stenografico 21 dicembre 2010 Gelmini pretende di fare, di riformare l’universitasenza adeguati investimenti che, esaltando il merito, diano la possibilita agli studenti meritevoli e anche a chi non ha le risorse di proseguire gli studi. Dopo aver provato a camuffare i tagli del comparto cultura, delle fondazioni liriche, della scuola pubblica, del sostegno al patrimonio culturale, ora questa riforma celebra il de profundis anche dell’universita. Considerare la ricerca come un utile ornamento dimostra la volonta di tagliare il futuro dei nostri giovani e quindi del Paese Oggi blindate questo provvedimento, come state blindando i palazzi del potere da una contestazione legittima, che i gesti di un manipolo di violenti non puosminuire. Noi dell’Italia dei Valori ci batteremo affinche´ questa riforma sia cancellata al piupresto. Con l’emendamento 2.21 si chiede di inserire, dopo le parole «risulti eletto»,

faccia presente alla senatrice Incostante che, a sua volta, lo farapresente, diligentemente, ai Segretari.

Vogliamo controllare, per favore? Controlliamo da una parte e dall’altra,

1, lettera d), sostituire le parole: «un unico mandato di sei anni, non rinnovabile», con le seguenti:

anche l’esito del suo operato, di rinnovarlo una sola volta, rispettando quindi la stessa durata di sei anni oggi prevista, ma permettendo una valutazione in piu, alla quale possa seguire un’eventuale rielezione. rielezione. Vogliamo altresı dire che l’Italia dei Valori ritiene il provvedimento un inutile braccio di ferro che il Governo sta imponendo al Parlamento e al Paese, pur non rappresentando la maggioranza degli italiani. Un vero eproprio atto di forza che il centrodestra, incurante del clima di particolare tensione che inquina la riforma, causato causato anche dall’arroganza del ministro Gelmini e della sua coalizione, che non hanno inteso ascoltare ne´ gli studenti, ne´ i ricercatori, ne´ tutti i precari che vengono sacrificati da una legge sbagliata, sta portando avanti. sta massacrando la ricerca e l’universita pubblica, che efuori da ogni logica e che va contro l’interesse del Paese. Noi dell’Italia dei Valori pensiamo che non si puo

studi. Dopo aver provato a camuffare i tagli del comparto cultura, delle fondazioni liriche, della scuola pubblica, del sostegno al patrimonio culturale, ora questa riforma celebra il de profundis anche dell’universita. Considerare la ricerca come un utile ornamento dimostra la volonta di tagliare il futuro dei nostri giovani e quindi del Paese Dimentico che del Paese a voi non interessa molto, visto quello che avete fatto fino ad oggi: solo leggi ad personam, e lo abbiamo visto, l’hanno visto anche parecchi elettori che dalla vostra parte stanno passando ad un altro tipo di ragionamento. (Commenti dal Gruppo LNP). Forse, quello di un Paese piu responsabile e di un Governo che pensa al Paese e non ad una persona sola. Oggi state blindando questo provvedimento, come state cercando di blindare i palazzi del potere da una contestazione legittima, che i gesti di un manipolo di violenti non puosminuire. Noi combattiamo questi violenti, signor Ministro, ma lei non deve sminuire ne´ la ricerca, ne´ i lavoratori, ne´ tanto meno chi nel comparto scuola vuole andare avanti a testa alta. Lei quella testa la vuole mozzare. L’Italia dei Valori si battera nel Paese affinche´ questa riforma sia cancellata il piu` presto possibile. Ma non solo questa riforma.

noi, invece, non siamo cosı soddisfatti e preferiremmo ritornare al testo del Senato che prevedeva un massimo di due mandati per non piudi otto anni. Noi crediamo che sei anni di mandato per un rettore siano troppi e che il mandato possa diventare troppo lungo, e crediamo quindi che un testo nel quale si preveda che dopo il primo mandato si possa

alle opposizioni, qualora le vogliano usare, di ottenere anche una dilazione dei tempi che qualche volta, evidentemente, esprime un dissenso che usa tutti gli strumenti regolamentari. (Applausi

Il metodo proposto serve a limitare lo strapotere del consiglio di amministrazione il quale, se da un lato avrail meritorio compito di tagliare corsi inutili, dall’altro rischia di divenire, come purtroppo grazie a questa riforma sara, il vero dominus delle universita`.

le seguenti parole: obiettare all’utilizzazione dell’espressione «codice etico», che purtroppo estata anche introdotta dalla Camera nel comma 4 dell’articolo 2. Essendo un liberale, non riesco a comprendere bene che cosa significhi «codice etico»: comprendo invece bene cosa significa «codice deontologico», e questa era l’espressione approvata dal Senato.

effettivamente rimossa l’espressione «codice etico» dal testo e sostituita con l’espressione piu corretta: «codice deontologico».

abbia colto l’occasione di questo emendamento per dimostrare quanto il lavoro fatto dalla Camera sia stato peggiorativo, e non solo in questo contesto in questo contesto del disegno di legge, ma complessivamente, come anche il relatore della prima lettura, senatore Valditara, ha avuto modo di rappresentare ampiamente in Commissione

Questa non euna leggina; voi l’avete chiamata riforma epocale ma, mi chiedo: puo una riforma, definita dal Governo «epocale», essere soffocata da ragioni di tempo e portare il Presidente della Commissione istruzione pubblica ad invocare il Governo affinche´ successivamente sia cambiata? Come si fa a non cogliere

Penso peroche i contenuti siano piu importanti dei modi, signora Ministro: lei ha sentito l’invocazione e l’auspicio del presidente Possa, segno che questo testo einadeguato

purtroppo, la Camera ha inserito tale dizione, che effettivamente non e adeguata. In questo contesto si chiede che si tenga conto del codice che avremmo voluto deontologico… ASCIUTTI

nello stesso codice (deontologico o etico) deve essere contenuto un principio, un criterio che presieda al meccanismo della presentazione delle candidature e dell’individuazione degli esterni.

– origine nazionale o sociale». L’emendamento in esame e volto sostanzialmente all’inserimento di un principio ispiratore importante tanto quanto quello delle pari opportunita:

prevedere che la nomina di detti membri sia ispirata anche e soprattutto ai principi di non discriminazione per qualsivoglia motivo. Per questo, chiediamo di rettificare il refuso contenuto

pur non rappresentando la maggioranza degli italiani, un inutile braccio di ferro: un vero e proprio atto di forza del centrodestra, incurante del clima di particolare tensione che l’iniqua riforma sta generando, clima causato dall’arroganza del ministro Gelmini e della sua coalizione, che non hanno inteso ascoltare ne´ gli studenti, ne´ i ricercatori, ne´ i precari, che vengono sacrificati da una legge sbagliata.

di riformare l’universita senza adeguati finanziamenti che, esaltando il merito, diano la possibilitaa tutti gli studenti meritevoli, anche a coloro che non hanno le risorse, di proseguire gli studi. Dopo aver provato a camuffare i tagli del comparto cultura, delle fondazioni liriche, della scuola pubblica e del sostegno al patrimonio culturale, ora questa riforma celebra il de profundis, anche e purtroppo, Considerare la ricerca come un inutile ornamento dimostra la volontadi tagliare il futuro dei nostri giovani, quindi del nostro state blindando questo provvedimento, come state cercando di blindare i palazzi del potere da una contestazione legittima, che i gesti di un manipolo di violenti non puosminuire.

Colleghi, e` presente in tribuna una delegazione di imprenditori cinesi del settore energetico. A loro va il saluto dell’Assemblea.

Il Senato non approva.

votare ognuno dal proprio posto

Non c’ealcun riferimento alla sua persona: perche´ ci dovrebbe essere? Ma certamente lei ha votato ripetutamente per un collega che si trovava altrove. A me chi lo dice? Perche´ mi impedisce di parlare? Chi me lo dice che il suo collega e altrove? Chi me lo indica? Io ho appreso che il collega era altrove nel momento in cui si esollevato il problema: lei me l’ha detto, io ne prendo atto la ringrazio, ma a me non lo diceva nessuno che il collega Marino era in giro per l’Aula. Al limite, potevo accorgermene se era lı vicino: ma lei, per caso, pensa che dovevo inseguirlo?

Presidente, sull’emendamento 2.118, prima firmataria la senatrice Vittoria Franco, chiedo ai colleghi di sostenere la mia richiesta per effettuare la votazione elettronica.

Appena me li diranno, li faremo.

Segretario Baio, tolga tutte le tessere di chi non e` presente sul posto.

Mi piacerebbe che i colleghi che non hanno potuto seguire da vicino i lavori per realizzare il testo di questa non riforma sapessero cosa votiamo. Alla Camera, incredibilmente superando il ministro Tremonti e il ministro Gelmini, i nostri colleghi hanno specificato, proprio ladove si dovrebbe valorizzare l’internazionalizzazione,

conterete quante volte e ripetuta la frase: «senza nuovi o maggiori oneri». E[]una riforma che si fa senza oneri, perche´ si conclude cosı anche l’ultimo comma dell’ultimo articolo.

Rimane il rimpianto, mio personale, in questa legislatura, di non aver potuto partecipare alla realizzazione di una riforma radicale, perche´ non equesta quella di cui l’universita italiana ha bisogno.

che nella riforma Gelmini eriferito al Ministro e al Ministero, nella riforma del PD e sempre attribuito agli statuti, che sono la Carta costituzionale dell’autonomia universitaria. Abbiamo predisposto un articolo intero per stabilire come deve avvenire il finanziamento sistematico, anno per anno, affinche´ i piani pluriennali siano noti a priori: abbiamo dato questa responsabilitaall’universita.

sapendo che dovevamo affidare il nostro tempo, la nostra intelligenza e la nostra passione a favore dei giovani e del sapere. La societa della conoscenza non viene arricchita con questo disegno di legge. Quando saraapprovato, sara piupovera la ricerca, piu povera l’universita. Questo emendamento e esattamente l’epitaffio, «senza nuovi oneri a carico dello Stato».

(FLI). Signor Presidente, voteroa favore di questo emendamento non per il contenuto in se´, ma per il fatto che solleva uno dei punti fondamentali di qualunque riforma dell’universita e della ricerca.

Il punto fondamentale e che all’universitae alla ricerca non vengono date risorse ne´ scarse ne´ abbondanti, ma semplicemente disperse a pioggia. Per non annoiare troppo i colleghi, ricordo solo che – per quello che risulta agli atti – in Italia sono 374 le sedi universitarie, le sedi universitarie, nelle quali risultano in media tre studenti per ogni docente. Allora il tema, cari colleghi della maggioranza e dell’opposizione, non e

20 centri di eccellenza ai quali concedere l’autonomia di fare la formazione piualta, che e quella dei dottorati di ricerca. di ricerca. La mia generazione ha aspettato 25 anni per avere i dottorati di ricerca in Italia: dovevamo andare all’estero per fare il dottorato di ricerca. Quando li abbiamo realizzati, li abbiamo dispersi in 1.000 cose che

del coraggio politico di valutare l’enormita delle risorse che spendiamo per l’universitae per la ricerca rispetto

i miei figli, i figli dei ricchi, possono accedere ai livelli alti di istruzione, ma i figli dei poveri sono esclusi in partenza. Questa ela vera sfida politica, che non si risolve certo

perche´ e troppo poco, perche´ bisognerebbe fare di piu. Ma di fronte a questo troppo poco c’e la rincorsa ad andare sui tetti per farsi riprendere dalle televisioni e stringere la mano a certe organizzazioni, non distinguendo tra l’interesse vero e legittimo degli studenti e dei docenti seri e quello di quanti in realtabivaccano dentro le nostre universita. Dopo di che fa un provvedimento per il rientro dei cervelli, pensando che con 200 euro al mese di sconto dell’IRPEF i nostri migliori ricercatori rientrino in Italia:

Signor Presidente, solo una battuta: molti degli argomenti usati dal senatore Baldassarri sono assolutamente condivisi da quella che lui ha definito la «sua maggioranza». Spero non sia una reminiscenza del passato, ma piuttosto, visto che stiamo parlando di legge universitaria, mi auguro che il senatore Baldassarri abbia studiato tanto e quindi si trovi avanti sul programma del suo Gruppo al Senato. (Applausi Signor Presidente, ho ascoltato con crescente incredulitala perorazione del senatore Baldassarri. parlasse per appoggiare le motivazioni nobili e ben argomentate della senatrice Garavaglia, su un tema che viene perennemente ripetuto qua: la riforma senza soldi.

A mano a mano che andava avanti a parlare, sembrava pero che cambiasse progressivamente opinione e, per slittamenti successivi, earrivato alla fine a dire quasi il contrario di quello che ha detto detto il senatore Baldassarri. Individuare gli studenti e i ricercatori in agitazione come un manipolo di scalmanati che bivaccano e veramente terribile. Colleghi, mi sembra che se si ragiona in questa maniera, in quest’Aula si perda materialmente la capacitadi apprezzare il contributo soggettivo il contributo soggettivo che le forze attive della societa danno. Il fatto che alcuni ricercatori siano saliti sul tetto non significa che non pubblichino articoli, che non facciano lezione, che non si impegnino, certe volte allo spasimo, e spesso con stipendi inverosimili, e qualche volta gratuitamente, per determinare la formazione dei loro studenti. Semplicemente, aggiungono ad un carico personale di attivitanell’universita anche l’impegno per sollecitare l’opinione pubblica, per far capire che cosa succede. Se il ricercatore sale sul tetto, cari colleghi, non euna manifestazione di stravaganza: e perche´ l’opinione pubblica, la societae quest’Aula alla fine sono sorde, non ascoltano, non sentono, non intendono.

del Partito Democratico, almeno quelli che hanno pensato nella direzione che adesso diro, farebbero bene a ritornare sulle loro intenzioni. Mi sembra infatti davvero difficile pensare che il Partito Democratico, che ha condotto una lotta seria su questa legge,

il cosiddetto terzo polo. Forse farebbero bene a ripensare questa soluzione, perche´ sul terreno fondamentale della edificazione di una scuola e di una universita` ci sono davvero due pareri opposti e su questo bisogna bisogna riflettere. Lo dico da amico, non per fare una polemica cattiva: lo dico perche´ questo mi pare nel futuro un argomento da prendere molto sul serio.

]un po’ il paradosso del dibattito in libertasulla riforma universitaria. Ma a parte questa considerazione e valutazione, credo che le riflessioni che ha fatto il senatore Baldassarri siano provocazioni culturalmente ed intellettualmente oneste e corrette che ci dicono come siamo dentro un percorso, nel quale abbiamo il dovere di stabilire un punto fermo

che per noi e un dato di partenza e non un punto di arrivo. Infatti vorremmo che il dibattito parlamentare, anche attraverso la capacitadi dare dignita alle proposte contenute negli ordini del giorno, indichi un percorso da seguire rispetto al quale il Governo e qualsiasi maggioranza hanno il dovere del dialogo e del confronto, perche´ ci troviamo – altrimenti non diamo dignitaal lavoro che si compie – di fronte ad una riforma di sistema ad una riforma di sistema che riguarda la destra, la sinistra ed il centro, e non l’attualita del Governo, ma il futuro; deve esprimere una visione. Per questo, mi auguro che interventi come quelli della senatrice Garavaglia e del professore e senatore Baldassarri servano a stabilire questo clima di dialogo e di confronto alto, perche´ di questo abbiamo necessita` e bisogno, perche´ di questo ha bisogno il Parlamento per qualificarsi sul terreno di una riforma fondamentale.

Il senatore Quagliariello si e compiaciuto poco fa per un’espressione del senatore Baldassarri, che ha dichiarato: «la nostra maggioranza». Sarei piuprudente se fossi il senatore Quagliariello, perche´ ho visto troppe volte, in queste ultime settimane, che quel che la mattina e maggioranza il pomeriggio e` diventata opposizione, e viceversa. Quindi sarei molto prudente,

l’intervento della senatrice Garavaglia, e anche del collega di Futuro e Liberta– che qui e stato sottolineato anche da quanto ha detto poco fa il senatore Viespoli – ha sollecitato certamente un intervento fuori luogo del senatore Pardi rispetto a quello che puoessere il volto del terzo polo, la sua disponibilita nei confronti di una legge ordinamentale cosıimportante e significativa per il futuro dell’universita ed anche per un approccio diverso all’universitastessa nel nostro Paese e di cui c’e assolutamente bisogno. Vorrei ricordare al senatore Pardi che siamo in un cammino, come terzo polo, che vedraun confronto serio ed approfondito su tutte le questioni, in modo particolare su quello della cultura, della scuola e dell’universita.

passata stesura di questo testo al Senato espresso un voto contrario che riguardava in modo particolare la mancata copertura finanziaria. La nostra attenzione, senatore Pardi, alla Costituzione ed ai problemi della scuola e dell’universita eprofonda e nel tempo e stata sempre costante. Una vicinanza agli studenti prima che agli insegnanti, una vicinanza complessiva a tutto il sistema universitario che ha bisogno assolutamente di essere rinnovato, cambiato e adeguato alle esigenze della modernitae dell’internazionalizzazione della stessa cultura e degli stessi strumenti con cui la cultura viene prodotta. Pertanto – ripeto abbiamo avuto questa posizione e stiamo attenti sia a quanto sta facendo tutta l’opposizione, sia soprattutto a quanto puo essere oggi dimostrato dal Governo come opportunitae disponibilita ad accogliere le nostre istanze. Non ci faremo assolutamente lusingare, come non abbiamo fatto ieri,

e resteranno tali nella difesa non di interessi partitocratici o di parte, ma nell’interesse dell’universita` italiana, dei giovani, che hanno diritto a un futuro migliore, e anche di chi vi lavora per il bene del Paese.

Signor Presidente, lei eandato cosı veloce che non sono riuscito prima a farmi vedere quando ho chiesto la parola, ma la prendo adesso, non solo per sostenere convintamente questo emendamento 2.135, ma anche per esprimere il disappunto sulla non ammissibilitadell’emendamento 2.309, che mi sembrava

che ancora non e stato nominato il consiglio direttivo, benche´ le procedure di presentazione delle candidature siano state chiuse il 20 settembre. A tre mesi di distanza,

negli Stati Uniti, l’Educational Testing Service, che e` un’agenzia privata, una delle tante che valutano gli studenti universitari, dispone di 1.500 dipendenti.

Tutto questo non c’e, il che vuol dire che tale riforma, basata sulla valutazione, non potraentrare in vigore se non tra moltissimi anni, quando sara costituito l’ANVUR, sarastato finanziato e avra sperimentato le procedure e finalmente sarain grado di valutare. Mi dispiace che l’emendamento 2.309 sia stato dichiarato inammissibile, ma soprattutto dispiace che questo cardine, questa terza gamba del sistema universitario ancora non esista, se non nei piani e nella immaginazione dei dirigenti del Ministero. Forse sono

radicalmente contrario al progetto di legge, tanto evero che adesso vuole che siano approvati degli ordini del giorno che diranno in che modo vada riformata questa riforma.

ha tratto delle conclusioni che sono l’opposto di quelle che io avevo tratto. Per chiarezza, su questo provvedimento do un giudizio positivo. La mia critica eche e troppo poco rispetto al tanto che bisognera` fare.

onorevole Sottosegretario, colleghe e colleghi, questo emendamento, che per alcuni versi assomiglia a quello illustrato cosıefficacemente dalla collega Garavaglia, e un emendamento che, in verita– vi prego di prestare attenzione sul punto – disvela il senso profondo, in un certo senso, il sottotesto di questa articolata stesura di norme (come sapete, sono 173 che diventano 500 in un corpo normativo sull’universita di 1.500 giaesistenti: dunque, un pasticcio burocratico incredibile), quindi la verita dei fatti. Ci ammoniva Aghata Christie che spesso il diavolo si incarna nei particolari ed il colpevole lascia delle tracce. Ebbene, la frase «senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica»,

Si poggia, come una palafitta barocca, ma di plastica, sul niente, su una sorta di territorio melmoso. Tale emendamento e la vera realtadi questo testo. che questo punto sia chiarito anche nel voto. Se non si accoglie questo emendamento, implicitamente si accoglie la menzogna di questo testo, che apparentemente euna riforma, ma in realta euna controriforma.

d’improvviso la necessitadi rendere conto ai colleghi del motivo per cui presentiamo gli emendamenti, altrimenti sembrerebbe davvero un fatto curioso presentarli. Comunque, ogni volta che ho parlato, credo si sia capito che non era un fatto ostruzionistico per perdere tempo. Il comma 11

esame alla fine la comunita accademica saraquella che conta di meno, perche´ non puo autoregolarsi attraverso uno statuto che garantisca l’ultimo comma dell’articolo 33 della Costituzione in quanto tutto e` precisato, anche troppo, quasi come in un regolamento, in questo disegno di legge. (Applausi dei

in questa materia. Il Fondo per il merito attiene alle opportunitadi percorso e di successo formativo degli studenti. Quindi, siamo pienamente all’interno della competenza, da un lato in termini di diritto lo studio, dall’altro di istruzione.

della Conferenza Stato-Regioni, laddove sono da definire i criteri per la gestione di questo fondo e anche la gestione del fondo stesso.

Basti pensare che rimanda essenzialmente a contribuzioni private, anche da parte di fondazioni, e non da alcuna certezza.

d’accordo con l’istituzione del Fondo per il merito, ma non ci si puo limitare soltanto a proclami che poi non hanno alcuna ricaduta concreta nella realta. realta. Proponiamo anzitutto che il Fondo per il merito sia esteso a coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca

deve o vuole studiare in una universita, puoquesta famiglia sostenerlo integralmente negli studi? E[ ]questa la domanda che ci dobbiamo porre.

Non si tratta soltanto di una questione astratta di giustizia, di uguaglianza, ma anche di opportunita, al fine di non disperdere talenti e risorse umane nel nostro Paese. poi l’erogazione dei premi di studio, finalizzata alla copertura di oneri derivanti dall’iscrizione e dalla frequenza di universita pubbliche per studenti al di sotto di una soglia di reddito.

si prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro a decorrere dal 2011 per il funzionamento del Fondo per il merito.

eche le risorse diventano sostanza e certezza di riforma. Una riforma non puo adagiarsi sulla logica del «se ci sono le risorse»,

Ecco la ragione per cui noi abbiamo riscritto un articolo che disciplina il Fondo per il merito, che euna misura positiva a cui noi crediamo, – proprio perche´ ci crediamo – vogliamo che esso sia una certezza, una garanzia, e non soltanto un flatus vocis per poter fare un po’ di propaganda.

a prescindere pero dal diritto allo studio. Al contrario noi puntiamo molto sul diritto allo studio, che si realizza attraverso il riconoscimento del merito alle persone

Pero qui non si parla di giustizia, non si danno gli strumenti per realizzare una societapiu giusta perche´ non si seleziona anche in base al reddito, ma solo in base al merito. In altri termini, si schiacciano le persone

gli studenti vengano selezionati in base al merito e al reddito. Stiamo vivendo in questi mesi e in questi ultimissimi anni in una societa preda e vittima della crisi economica, nella quale esiste uno squilibrio totale nella distribuzione della ricchezza. E[]cresciuta la poverta. Il destino dei figli esempre piu definito dalla posizione sociale e dalle risorse a disposizione della famiglia di provenienza.

battaglia per il merito, ma puntiamo molto al riconoscere la possibilitadella mobilita sociale. Attribuiamo molta importanza ai nostri emendamenti che introducono questo elemento e mi auguro davvero che l’Aula almeno questo possa approvarlo.

quanto giaillustrato dalla senatrice Vittoria Franco relativamente alla nostra visione di accoglimento e di approvazione del Fondo per il merito, ma nell’ottica di un collegamento, nella gestione di questo Fondo, dei criteri relativi all’eccellenza con quelli relativi al reddito. Quindi, proponiamo di assegnare i premi di studio in concomitanza dell’inizio dell’anno accademico. Capiamo tutti quanto sia importante, per chi ha condizioni di reddito non adeguate,

ad una soglia di reddito che annualmente verra parametrata dal Ministero. E[] evidente che non si tratta delle soglie di reddito molto basse, le quali danno accesso al diritto allo studio, bensı di quelle soglie comunque indispensabili per non erogare i premi di studio a quei ragazzi le cui famiglie hanno condizioni economiche di assoluto agio. Sappiamo infatti che nell’universitaesiste

con quelli relativi al diritto allo studio, ma deve essere tenuto in considerazione. Quindi, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, chiedo di prestare attenzione su questo punto, che e assolutamente dirimente per la visione alla quale vogliamo improntare l’universita, attribuendo ad essa quel valore di percorso che favorisce la mobilita sociale, assolutamente fondamentale per il futuro di tanti giovani e dello stesso nostro Paese.

votazione). Il Senato non approva.

che appartiene ad una famiglia con un miliardo di reddito annuo viene trattato esattamente come il figlio di una famiglia che non puoarrivare alla fine del mese.

dei giovani prende le borse di studio, ma mancano le borse di studio per i giovani meritevoli e bisognosi. E[]una cosa gravissima: per questo chiedo che questi emendamenti vengano votati,

premialita del merito. Stabilendosi infatti che sono esclusi dall’obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica con il massimo dei voti,

suo complesso eun po’ troppo accentuato sulla demagogia del merito, e parla una persona che per cultura ha sempre sostenuto il merito, per quanto esso effettivamente vale e puo produrre in termini positivi.

pregherei davvero i colleghi di ascoltare. Alla lettera o) del comma 3 di questo articolo 4, si dice che, nell’ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, si riserva la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle universitadella Regione in cui risultano residenti. L’ho letto due volte perche´ pensavo vi fosse un refuso,

cosa che e teorizzata in tutto il disegno di legge. Ma, ministro Gelmini, evidentemente lei ha voluto accettare un emendamento, immagino, leghista – dato che di qualsiasi cosa si parli, i leghisti chiedono la riserva per i residenti

siano i migliori. Siccome costruiamo un fondo apposito per i migliori, capaci e, meritevoli, e il primo obiettivo del fondo e mandarli all’estero,

Si incoraggia cioela residenzialita in un disegno di legge che econtro le gemmazioni (che peraltro ha fatto il ministro Moratti, come lei ricordera bene); stabilisce che i centri di eccellenza devono essere pochi,

poi chiedere la riserva per quelli che frequentano, come direbbero i miei amici della Lega, a casa loro. Noi pensiamo che questo

all’articolo 4, comma 3, sono elencati i criteri con cui dovranno essere distribuiti; premi di studio e, buoni di studio. L’ultimo di questi criteri, alla lettera o), introdotto dalla Camera, prevede che vi sia una programmazione di tipo regionale degli accessi alle borse di studio.

delle finanze, e` alimentato con: a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, societa, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalita del fondo, a specifici usi; usi. L’emendamento evolto alla soppressione di un periodo il quale riguarda le modalita operative con le quali lo Stato, cosı` viene indicato,

rinviare alle calende greche qualsiasi altro provvedimento successivo all’approvazione della riforma. Chiediamo pertanto che venga un po’ ridimensionato il potere del Ministro dell’economia. Signor Presidente, anche noi, come Italia dei Valori, chiediamo con l’emendamento 4.40 di eliminare la previsione secondo la quale sia sempre e comunque il Ministero dell’economia a gestire l’istruzione, l’universitae la ricerca. Il fondo di cui al presente articolo deve essere gestito, lo ribadiamo anche noi, dal Ministero dell’istruzione, dell’universita e della ricerca e non dal ministro Tremonti, il quale ha giacommissariato il ministro Gelmini sull’istruzione primaria e secondaria. Il ministro Tremonti, che purtroppo e da tempo che non vediamo qui in Aula, non puopensare di riformare l’universita senza adeguati finanziamenti che, esaltando il merito, diano la possibilitaa tutti gli studenti meritevoli, anche a coloro che non hanno le risorse, di proseguire gli studi. Dopo i tagli lineari al comparto

votazione). Il Senato non approva.

parere favorevole.

Presidente, vorrei illustrare brevemente l’emendamento 5.4 che riguarda la realizzazione di azioni di orientamento per gli studenti delle scuole superiori, anche al fine di incentivare le iscrizioni nelle facoltascientifiche. Il presidente Possa sa quanto quanto abbiamo discusso di questo tema e dell’opportunita dell’incentivazione di queste iscrizioni. Il non accoglimento di questo emendamento mi sembrerebbe davvero assai incongruo. Ne sottolineo l’importanza con questa mia illustrazione.

cosıcome previsto dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), e devono essere protesi a garantire il livello di istruzione superiore, che non puo avere ostacoli di ordine sociale.

e la responsabilita la si esercita semplicemente attraverso la premialitain base alla valutazione. Con l’emendamento 5.311 proponiamo che ci sia una quota crescente

venga destinata a missioni scientifiche o di ricerca di interesse nazionale. Ci sembra un buon modo per valutare davvero il lavoro delle universita` e quindi per distribuire i fondi in base davvero al merito, in questo caso.

e di fronte alla sfiducia che manifestano verso la classe dirigente di questo Paese, il nostro compito sicuramente equello di interrogarci e di comprendere, ma ancor piu di dare risposte concrete,

alloggi che servono agli studenti meno abbienti, a quelli che per seguire i propri interessi e per sviluppare le proprie capacitavanno lontano dalle loro case, per spezzare un sistema speculativo presente in molte citta italiane nei confronti degli studenti e delle loro famiglie attraverso l’evasione fiscale e gli affitti in nero, e per dare un luogo di socialitae di tranquillita agli studenti. Qualcuno di voi ha detto che vuole dialogare con il movimento degli studenti. C’eun modo per farlo: approvate questo emendamento. Solo la concretezza delle nostre risposte puo dare risposta alla speranza dei troppi che ancora non ce l’hanno. Dimostrate, votando a favore di questo emendamento, di non avere come unica risposta il ricorso ai DASPO.

credo che debba essere un tratto distintivo di una politica di sensibilita` che il Governo deve saper dimostrare. Come nella valutazione non ci possono essere criteri generalizzati a prescindere dal contesto, dalla persona in se´, e dalla sua storia culturale, oltre che umana, cosı, nel definire questi livelli essenziali, non possiamo prescindere da diversita che vanno considerate non soltanto come elementi ostativi, ma anche come opportunitache dobbiamo saper difendere nel loro valore di diversita. Chiedo al Governo un atto di sensibilitae di ripensare la possibilita

era stato discusso in Aula riguardo a un emendamento che, in riferimento ai portatori di disabilita, tiene conto appunto della loro disabilitaper definire i livelli di prestazioni essenziali.

non si puoprevedere il livello delle prestazioni essenziali a prescindere da diversita che vanno, invece, accolte nel loro valore e non nella loro potenzialitanegativa, cosı come si sottintende in questo emendamento.

L’emendamento egia stato votato, quindi non epossibile nessuna trasformazione in ordine del giorno. La senatrice Sbarbati ha posto un altro problema: di interpellare il Governo, che puo scegliere se vuole intervenire o meno, come sanno i colleghi, in qualunque momento. Lo decidera` il Governo se ritiene o non ritiene di intervenire.

Nell’ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni l’emendamento introduce ulteriori criteri per rendere effettivo tale diritto. Essi sono:

prevedere la realizzazione periodica di analisi della condizione studentesca e sui costi di mantenimento agli studi; approvare un Programma nazionale per il diritto allo studio; prevedere la realizzazione di un rapporto triennale sull’efficacia delle politiche di sostegno e dei servizi agli studenti;

garantire i servizi di assistenza sanitaria; promuovere lo sviluppo di un sistema di relazioni europee ed internazionali volto a migliorare la qualita` dei servizi del diritto allo studio universitario.

ci ha spiegato che eobbligatorio approvare questo provvedimento entro il 31 dicembre per non perdere risorse, soprattutto per il diritto allo studio degli studenti. Peccato che alla Camera il Governo ha fatto appiccicare a questo articolo 5 un comma 8, scritto in un pessimo italiano (per cui, Ministro, le suggerirei, magari consultando il ministro Brunetta, di disporre di collaboratori piu efficaci) introdotto da tre subordinate piuun anacoluto, che recita come

nell’impossibilita di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione eeffettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e allegata una relazione tecnica (…), che daconto della neutralita finanziaria» – cioe` a zero risorse – «del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti

Avremo prima, o tra quanti mesi, in merito al diritto allo studio per gli studenti che chiedono serieta di risposta (sono il 90 per cento, quelli che sfileranno pacificamente e hanno giasfilato pacificamente e quelli che stanno nelle aule), stanno nelle aule), i nuovi decreti senza risorse, o aspetteremo le risorse? E intanto, i decreti attuativi faranno invecchiare e diventare inutile questa legge? Ci dia questa risposta, perche´ e importante per gli studenti.

Per quanto attiene al diritto allo studio, come lei ben sa, nel miliardo di euro stanziato per l’universita, 100 milioni sono destinati al diritto allo studio, i quali, unitamente ai 25 giapresenti, rendono la cifra

per allineare la cifra stanziata per il diritto allo studio quest’anno sull’anno passato. Per quanto concerne il riferimento al rischio di perdere risorse, abbiamo giadetto e confermiamo, riguarda la necessita di bandire concorsi per promuovere i ricercatori, fra gli altri, al rango di professore associato; riguarda i 120 milioni di euro su base

bloccati dalla finanziaria. Queste sono le notizie che le dovevo fornire. Per quanto riguarda i decreti attuativi, ci stiamo gia lavorando e, in particolare,

Se comprendo bene, visto che il Piano per il Sud si alimenta di fondi strutturali e di fondi FAS, voi ovviamente utilizzerete i fondi destinati alle politiche di coesione per colmare un vuoto di bilancio sulle politiche ordinarie del suo Ministero. Mi pare la giusta filosofia per spiegare che il Piano per il Sud e soltanto una toppa e non ha alcun valore strategico. Usate i soldi destinati a cose ben diverse per colmare i tagli di bilancio che operate sul settore della scuola e della universita. Va bene cosı.

ad ogni frase e ad ogni periodo di questo disegno di legge il ritornello, di cui voi avete giaabbondantemente abusato, che tutto questo avviene senza oneri, cioe con i fichi secchi.

come si merita di sentirsi dire il presidente Possa, che la verita si conviene agli uomini onesti, perche´ gianell’articolo 4, alla lettera o), aveva detto: e cosınon cosınon precedentemente spiegato il contenuto di questo comma, che forse non sara mai attuato. Ecco, euna bella verita, perche´ in molte parti questa legge non saraattuata. Vicino al ministro Gelmini siede, opportunamente, il ministro Calderoli, perche´ qui si tratta di sapere, come nei LEP precedentemente discussi, quando si fa riferimento ad una delega per decreti legislativi, se si possa o meno contare su un bilancio. Ci siamo sentiti dire in quest’Aula dal ministro Tremonti che non poteva quantificare i decreti a valle della legge quadro sul federalismo. Qui e esattamente questo: «E nella impossibilitadi procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione e effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi». Poiche´ per ora, contrariamente al disegno di legge presentato dal Partito Democratico, collega Valditara (che all’articolo 1 decideva una volta per sempre come ecostituito il fondo di funzionamento ordinario, come ogni anno puo essere integrato dall’indice di inflazione, e quindi c’era la garanzia sui piani pluriennali e sui decreti legislativi), il disegno di legge in esame non ha il finanziamento e la modalita` di finanziamento, e dice che i decreti legislativi saranno finanziati. Ma quando? Non ci saranno decreti legislativi! Concludo come ha concluso il presidente Possa sulla lettera o) dell’articolo 4.

in modo efficace i colleghi Rusconi e Garavaglia. Hanno toccato il merito e quindi forse non vale insistervi. Approfitto di questo breve momento per sostenere che con questo con questo comma, gli estensori della legge hanno perso una occasione occasione per evitare di fare della cattiva prosa. La scrittura di questo testo e letteralmente infame,

Lei con correttezza ci ha detto prima le cifre e, quindi, ci ha confermato che, pur aggiungendo i 100 milioni,

Ministro, si ribelli a Tremonti: faccia sentire piu forte la sua voce nel Governo, perche´ l’Europa che conta va in un’altra direzione! Quella d’investire nell’innovazione, nella ricerca e nelle universita; quella di capire che la ripresa tedesca e anche frutto di questo investimento.

mettendo a disposizione 800 milioni di risparmio. Naturalmente siamo disponibili a controproposte. Come il Governo in altri momenti ha saputo trovare risparmi o proposte per l’Alitalia e per la prima casa, noi riteniamo che per il diritto allo studio le risorse si debbano e si possano trovare. Non si puo` venire in questa Aula e dire: riusciremo a dare solo 25 milioni in meno di quest’anno. Ci sembra una risposta inadeguata, signor Ministro. Investire in futuro e in merito, premiare gli studenti migliori vuol dire dare risposte diverse;

anche noi presentiamo delle prospettive di sostegno economico analoghe a quelle dei colleghi del Partito Democratico. E lo facciamo perche´ abbiamo la sensazione, purtroppo ampiamente provata, che il diritto allo studio sia in realtail grande ferito, il grande assente, il grande danneggiato di questa legge. Ci sono altri elementi di cui abbiamo discusso con energia, le contraddizioni e gli aspetti inaccettabili di questa legge, ma il mancato sostegno del diritto allo studio e forse fra tutti i danni il peggiore: l’assenza di risorse e di fondi a sostegno della possibilitadegli studenti di esercitarlo

sostegno per i meritevoli che concludono gli esami e il corso di laurea nei tempi previsti, sostegno per la realizzazione della propria qualitadi studiosi in formazione. Questo e un elemento che ein un certo senso il piu rilevatore della vuotezza intima e ontologica di questa legge.

il cui significato verrachiarito soltanto con i mezzi di attuazione; e di fronte all’incertezza di questi futuri mezzi di attuazione l’opacita del tutto si aggrava e si complica.

inerenti al diritto allo studio dovrebbe essere il compito essenziale di una legge sull’universita, invece tale aspetto viene a mancare completamente e non abbiamo possibilita noi, come minoranza in Aula, di interrompere questo pessimo costume che genera impossibilitadi risultati efficaci. Ci proviamo, presentiamo emendamenti, ma voi li bocciate e abbiamo di fronte a noi una sorta di abisso della formazione. Come si puo risolvere questa situazione? Non c’ealtra possibilita che la maggioranza si adatti ad una sorta di ravvedimento operoso, provi a prendere sul serio tali emendamenti e conceda ad essi l’appoggio che serve a determinare un risultato positivo.

balıa di se stessi, uno scandalo che si ripete senza che i responsabili siano chiamati a pagare, visto che sono stati assolti dal ministro Matteoli; oppure parlare di un altro grave scandalo, piu volte annunziato in questa Aula e raccontato in prima pagina domenica scorsa da Eugenio Scalfari. Affrontero` quest’ultimo tema, perche´ il maltempo passa, mentre i disastri provocati dai banchieri restano. Nell’atto di sindacato ispettivo 3-01814 segnalavo una notizia pubblicata dal «New York Times», secondo la quale il nocciolo duro della speculazione ecomposto dagli hedge funds, i fondi dedicati ad impieghi rischiosi che quando centrano l’obiettivo procurano elevati rendimenti, in tempi di bassi tassi d’interesse, e grave danni alla sovranita degli Stati. Stati. Il «New York Times» ha descritto pochi giorni fa il funzionamento di questa «cupola» ed ha anche indicato le banche che la compongono, ossia le banche di affari, che sono: Goldman Sachs (immancabile), Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, Barclays, Ubs e Credit Suisse. Ebbene, queste banche si riuniscono in